link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

non se ne può parlare ora; ne parleremo a fine seduta, secondo la prassi dei lavori parlamentari. Sull'ordine dei lavori si può intervenire, come sempre,

Ricorda che nella seduta pomeridiana del 29 luglio hanno avuto luogo l'illustrazione e la discussione delle mozioni.

culturali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, credo che nel corso del dibattito siano emersi, oltre a comprensibili critiche nei confronti del Governo da parte dell'opposizione, anche punti di vista comuni. Innanzi tutto, è emersa la condivisione di un punto fondamentale tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione e cioè che la cultura, soprattutto in un Paese come l'Italia, non è una spesa. La cultura in un Paese come l'Italia è un investimento,

non soltanto per il suo progresso economico e sociale ma anche per quanto riguarda il suo progresso civile e democratico. La cultura, La cultura, come ha ricordato il senatore Pittoni, è la nostra identità, è l'identità dell'Italia. Un Paese, perciò, che non investe nella cultura è un Paese che non ha un futuro. Certo, anche dai banchi dell'opposizione mi si potrebbe invitare, e lo comprendo, ad un maggiore coerenza, ad una maggiore determinazione nel difendere questi principi

ma voglio ricordare, per spirito di verità, che ciò di cui sto parlando è una tendenza storica del nostro Paese,

È esistita, credo, nel corso degli ultimi decenni della vita politica italiana, dal dopoguerra ad oggi, ad oggi, una sottovalutazione da parte delle classe dirigenti di questo Paese - intendendo per classi dirigenti non soltanto la classe politica, ma anche quella imprenditoriale ed il mondo culturale - dell'importanza che la cultura ha per lo sviluppo del nostro Paese. Credo che nessuno possa negare questo. Spendiamo da sempre poco, e meno di quanto non spendano tutti gli altri Paesi europei,

nonostante abbiamo compiti ben maggiori e più importanti circa la tutela del nostro patrimonio storico, che riguarda la nostra identità nazionale come popolo, rispetto agli altri Paesi.

Spendiamo male le poche risorse che abbiamo a disposizione, non le indirizziamo verso progetti qualificanti per il futuro del Paese, ma le disperdiamo molto spesso in mille rivoli. Inoltre, lo Stato interviene troppo e male nella cultura attraverso criteri burocratici, assistenzialistici e credo anche, cari colleghi, che meno lo Stato interviene nella cultura e più la cultura è libera, può esprimere appieno la propria creatività ed essere la massima espressione della libertà. Per questo credo che bisogna avere il coraggio di aprire ai privati.

lavoratori. Gli uomini di ingegno e cultura che lavorano nel mondo dello spettacolo e della cultura hanno la stessa dignità di tutti gli altri lavoratori.

attraverso una differenziazione di funzioni anche nell'erogazione dei fondi, tra manifestazioni di carattere locale e manifestazioni che riguardano istituzioni culturali nazionali che hanno anche un riflesso internazionale, come nel mondo della lirica.

deputati, com'è stato ricordato, è in discussione una riforma dello spettacolo dal vivo, con una possibilità di convergenza tra maggioranza e opposizione. Sono favorevole a questa riforma e spero che tutte le forze politiche possano continuare a sostenerla. Allo stesso modo sono

che è una prospettiva comune della maggioranza, ma anche dell'opposizione: era infatti un punto contenuto sia nel programma della maggioranza, che in quello dell'opposizione. Anche in questo caso sono favorevole alla riforma e la sosterrò nel dibattito in Commissione e in Aula, sperando che possa ottenere il consenso di tutto il Parlamento.

Quest'anno dobbiamo salvare il salvabile, la sopravvivenza stessa del mondo dello spettacolo: per questo era necessario un parziale reintegro del Fondo unico per lo spettacolo, per salvare il mondo dello spettacolo da una bancarotta, da un fallimento. lo ripeto - dobbiamo accingerci ad una profonda riforma di questo settore, a partire da quella delle fondazioni lirico-sinfoniche, che proporrò al prossimo Consiglio dei ministri di settembre. Voi sapete che al 31 dicembre 2008 le fondazioni lirico-sinfoniche hanno accumulato circa 300 milioni di euro di debiti, 300 milioni di euro di debiti, con un risultato di esercizio che nel quinquennio 2002-2007 ha registrato un passivo totale di circa 160 milioni di euro.

e nessuno sa più come uscire da queste difficoltà; i Sindaci stessi chiedono al Governo di intervenire, di fare qualcosa. E noi dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo intervenire, certamente, con riforme eque, giuste e condivisibili, ma dobbiamo fare qualcosa per interrompere questa spirale di debiti e di crisi che, ad un certo punto, può far saltare tutto, con rischi imprevedibili per la tenuta del sistema, e quindi per le sorti degli stessi lavoratori ai quali prima ho accennato. Certo, le fondazioni lirico-sinfoniche, come ricordava il senatore Possa - lo so bene - non sono soltanto i debiti,

Senatore, arrivo al punto e chiudo. Questa mattina si riunirà il Consiglio dei ministri il Presidente del Consiglio, come ha già dichiarato, annuncerà un parziale reintegro dei fondi del FUS che sarà, secondo me, sufficiente. Credo di aver rivolto all'opposizione parole di rispetto e non mi aspettavo una tale reazione. Come dicevo, il Presidente del Consiglio annuncerà stamattina al Consiglio dei ministri un parziale reintegro dei fondi del FUS che, secondo me e secondo gli uffici del Ministero, sarà sufficiente quest'anno a far fronte alle necessità. E io devo soltanto ringraziare,

a condizione che la stessa sia integrata del necessario riferimento alla riforma complessiva dei meccanismi di finanziamento e sostegno delle attività di spettacolo, nonché alla riforma del sistema lirico sinfonico a condizione che siano espunti dalla mozione alcuni riferimenti non accettabili: per esempio, la sottovalutazione dell'importanza dell'industria dei contenuti, o il riferimento ad una politica disinteressata al settore dello spettacolo da parte del Governo.

non solo a reintegrare il Fondo unico per lo spettacolo, ma anche a rivedere complessivamente i meccanismi di finanziamento dello spettacolo, tenendo conto di indici oggettivi, come l'affluenza del pubblico e la resa aziendale, nonché a riformare il settore lirico sinfonico, che versa in un profondissimo stato di crisi. Sulla mozione n.

ciò, peraltro, a condizione che vengano eliminate le seguenti espressioni contenute nel quarto periodo delle premesse: «ha di fatto messo in ginocchio il teatro, la musica e l'industria cinematografica italiana.

un chiarimento al signor Ministro. Mentre è accettabile la sua osservazione sull'inserimento delle riforme

la pregherei di riconsiderare questa sua richiesta. Mentre è accettabile l'evocazione delle riforme, il giudizio negativo è al di sotto di quello che ha dato lei.

e negli ultimi giorni in particolare, ha portato a prese di posizione, mobilitazioni ed assemblee per contrastare i tagli del Governo al Fondo unico per lo spettacolo per contrastare una politica che si sta dimostrando incredibilmente insensibile nei confronti di temi che dovrebbero a tutti stare a cuore. Per tali ragioni, signor Presidente, abbiamo chiesto come Gruppo dell'Italia dei Valori che prima della pausa estiva il Senato della Repubblica, attraverso la calendarizzazione delle mozioni, affrontasse con chiarezza un tema così delicato e di grande rilevanza ed esprimesse una volontà chiara e definitiva in favore del reintegro delle risorse che sono state sottratte al mondo dello spettacolo e al mondo della cultura, riportando il Fondo unico per lo spettacolo almeno ai livelli della legge finanziaria 2007. Negli ultimi giorni, signor Ministro, centinaia di artisti italiani e di lavoratori del mondo dello spettacolo, insieme a tantissimi rappresentanti di istituzioni culturali private e pubbliche del nostro Paese, del nostro Paese, hanno manifestato e sottoscritto un appello al Governo affinché provveda celermente, anche attraverso nuove regole al sostegno e allo sviluppo dello spettacolo italiano. Sempre in questi giorni anche il Capo dello Stato ha voluto far sentire la sua voce preoccupata, per sottolineare quanto la cultura e lo spettacolo debbano essere tenuti in considerazione nell'azione di Governo. Ancora una volta, signor Ministro,

Non è una novità per il nostro Paese, purtroppo. In Italia, il tema di fondo resta quello di una sostanziale debolezza e marginalità delle politiche culturali e di una subalternità di queste nei confronti delle politiche economiche e di bilancio. Mai però si era arrivati ad una situazione così grave da mettere seriamente in discussione la stessa sopravvivenza di tantissime istituzioni di spettacolo in tutta Italia. Mai si era arrivati ad una così ingiustificata riduzione delle risorse disponibili tale da vanificare il lavoro e le speranze di tutto il mondo dello spettacolo italiano, uno dei settori che hanno fatto grande il nostro Paese. Il bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali, a nostro avviso, è assolutamente fallimentare. Assistiamo giornalmente

per le sorti del mondo del teatro, della lirica, della musica, di chi lavora in questo settore, e ha affermato di confidare nella sensibilità del suo collega Tremonti. Signor Ministro, lei afferma di voler perseguire una politica di riforme che permetterà all'Italia di salvaguardare il patrimonio culturale. Dice, infine, di essere ben consapevole del fatto che questo settore ha saputo negli anni dare al Paese, anche in termini economici, molto di più di quanto non abbia ricevuto. Adesso vorremmo sapere se lei è davvero il Ministro per i beni culturali; noi riteniamo di sì! Non è stato forse il totale immobilismo del suo Ministero a paralizzare il settore in una indeterminatezza e in una attesa di interventi ed azioni annunciate di continuo, ma che finora non sono arrivate e che hanno determinato, insieme alla ingiustificata e gravissima riduzione delle risorse, una situazione di paralisi e di crisi del settore?

che hanno reso ricco questo Paese, e che, alla ripresa di settembre, molte di queste istituzioni saranno costrette a chiudere? La musica, l'opera, la prosa, il cinema, la danza hanno arricchito questo Paese. Le fondazioni lirico sinfoniche, le orchestre, i cori, le associazioni concertistiche e i teatri stabili di prosa, il grande mondo del cinema e il grande mondo della danza hanno offerto un contributo straordinario al livello culturale e all'economia del nostro Paese. È davvero incredibile che questo Governo faccia finta di non capire quale danno irreversibile stia determinando al nostro Paese

avrebbe potuto accogliere le nostre innumerevoli richieste in Commissione. Lei sa quante volte abbiamo richiesto la sua presenza in Commissione per condividere insieme a lei un percorso per una riforma vera e per affrontare temi così delicati: ma non è stato possibile. Lo ripeto: più volte,

di arte, dello straordinario patrimonio artistico del nostro Paese e dei tanti cittadini onesti che credono che si debba investire nella cultura e non spendere per essa. Nei mesi scorsi avevamo avviato un importante percorso all'interno della 7a Commissione permanente del Senato, approvando all'unanimità, tutti insieme, una risoluzione che dettava principi e linee guida per un progetto di riforma vero, al quale il Gruppo dell'Italia dei Valori avrebbe dato il proprio contributo e continua a volerlo offrire. Tutto ciò per l'interesse e per l'attenzione alla cultura e al mondo che gira intorno ad essa. Ma la disattenzione, l'assoluta inadeguatezza politica di questo Governo ogni giorno confermano le nostre preoccupazioni e le nostre perplessità, che per fortuna sono agli atti e nei resoconti delle Aule parlamentari. Bisogna cambiare e subito, prima che sia troppo tardi. Mentre negli altri Paesi europei le politiche culturali rappresentano per i Governi uno strumento importante di investimento e di crescita della collettività, in Italia questo non accade e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Da parte di questo Governo non vi è nessun interesse per le politiche culturali, che non sono considerate strumento per migliorare la qualità della vita delle nostre comunità e per investire sul futuro. La cosa è, purtroppo, in sintonia con la scarsa attenzione rivolta ai temi della scuola, dell'istruzione e della ricerca, che continuano ad essere residuali nei disegni di questo Governo, contribuendo così a delineare il quadro di un complessivo mancato investimento sui temi della cultura, della formazione e della ricerca. Il che, in questi mesi di drammatica crisi economico-finanziaria globale, stride fortemente non solo con le strategie adottate dei principali Governi europei, ma anche con 1'atteggiamento della nuova amministrazione americana, che dichiaratamente sta puntando sulla ricerca, sull'istruzione, sulla cultura e sulla innovazione per affrontare meglio la recessione internazionale. Deve ripartire una stagione in cui le politiche pubbliche devono assumere il tema della cultura come elemento centrale di attenzione per l'azione di governo: una nuova stagione. L'intervento pubblico nel settore della cultura, della musica lirica e sinfonica, della prosa, della danza, del cinema deve essere considerato un vero e proprio investimento e non una spesa improduttiva; lo diceva anche lei, signor Ministro. Al contrario, il nostro Paese, pur essendo depositario della parte più consistente del patrimonio culturale del mondo, è uno di quelli che investe meno in questo campo. In questo quadro generale di crisi siamo anche molto preoccupati per la sorte delle fondazioni lirico sinfoniche. L'opera lirica è ancora oggi uno dei prodotti culturali italiani di eccellenza nel mondo. È proprio intorno all'opera lirica che sono stati tramandati significati poetici, sociali, tradizioni artistiche ed artigianali ancora vive ed apprezzate. teatri d'opera italiani, le fondazioni lirico-sinfoniche, hanno avuto e hanno ancora oggi la funzione fondamentale di tramandare questa straordinaria tradizione e ricchezza del nostro Paese. I dati dimostrano che gli spettacoli e le attività delle fondazioni generano e, talvolta, sostengono in modo considerevole numerose iniziative economiche ed imprenditoriali ad esse collegate, direttamente ed indirettamente, sul territorio. Si pensi, ad esempio, al portato di queste iniziative sul turismo culturale, che dovrebbe costituire sempre di più una risorsa fondamentale per il nostro Paese. A tutto questo il Governo risponde con un taglio indiscriminato delle risorse che ha messo in crisi tutto il sistema. È appena il caso di ricordare che in atto ben tre fondazioni, signor Ministro, sono commissariate (il San Carlo di Napoli, il Carlo Felice di Genova e l'Opera di Roma) e una lo è stata fino a qualche mese fa (l'Arena di Verona): una situazione drammatica, mai verificatasi in passato. Peraltro, il venir meno dell'intervento dello Stato genera un effetto conseguente, non solo su quello delle Regioni e degli enti locali, le cui risorse sono state particolarmente ridotte dagli interventi del Governo, ma anche sull'impegno delle imprese che, nell'ultimo decennio, per la prima volta, sono state coinvolte a sostegno della gestione, con contributi, in qualche caso, significativi. Lo strumento delle fondazioni, seppur richieda interventi normativi che risolvano alcuni problemi messi in luce dall'applicazione delle norme e dall'esperienza di questi anni, ha tuttavia consentito il raggiungimento di importanti obiettivi di efficienza, di efficacia e di maggiore operatività gestionale. Molti dei problemi evidenziati nel dibattito più recente (sprechi, diseconomie, scarsa produttività del lavoro, insufficiente qualità artistica, limitato coinvolgimento dei privati, depauperamento del patrimonio), rispetto ai quali viene denunciato lo stato di crisi del settore, vanno approfonditi e, così come diceva lei, signor Ministro, verificati caso per caso, e comunque sono spesso la conseguenza proprio di una progressiva inadeguatezza delle risorse disponibili a causa delle continue oscillazioni del FUS e dei tagli che molte volte sono stati operati in in corso d'opera e in maniera indiscriminata. Il regime di costante incertezza rispetto alle risorse disponibili ha condizionato l'operatività delle fondazioni e anche molti risultati di gestione. Dunque va individuato uno strumento che ponga, intanto, le condizioni perché tutti abbiano, con il giusto anticipo, certezza delle risorse disponibili in un'ottica triennale. Noi crediamo che non vada dimenticato che il settore dello spettacolo è ad altissima specializzazione e con particolari specificità che lo rendono difficilmente omologabile ad altri comparti; ad altri comparti; che in esso lavorano migliaia di lavoratori che tramandano una tradizione che non ha pari nel mondo; che esso produce un indotto di grande importanza per l'intera economia del nostro Paese. Di tutto questo non si può non tenere correttamente

Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, la Lega Nord presenta la propria mozione per impegnare il Governo a modificare la gestione e la distribuzione, oggi accentrata, dei finanziamenti pubblici previsti dal FUS attraverso appositi strumenti normativi. Gli operatori dello spettacolo sono preoccupati dal fatto che lo Stato abbia sensibilmente diminuito la quota di finanziamento del FUS che sostiene enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante. Occorre ricordare che gli operatori del settore sono 200.000 e certamente è ragionevole la loro preoccupazione. E certamente ci auguriamo che il FUS venga incrementato, anche se ciò non basta. Se approfondiamo infatti il contesto dei finanziamenti al comparto dello spettacolo, ci accorgiamo che circa il 50 per cento dei fondi viene erogato dallo Stato, mentre la restante quota proviene ancora dallo Stato con finanziamenti speciali e dalle Regioni e dagli enti locali. Questo a significare che le Regioni e gli enti locali, pur in assenza di una legislazione nazionale *ad hoc*, hanno sviluppato una loro attività nel settore, prevedendo investimenti propri sul piano della progettazione, della promozione, della comunicazione e del sostegno alle diverse iniziative culturali del territorio, oltre che di connotazione nazionale ed internazionale. Alcune Regioni hanno anche sviluppato una legislazione propria in merito. Del resto, anche la Corte costituzionale, attraverso le sentenze nn. e 256 del luglio 2004, originate da una questione posta dalla Regione Toscana circa il conflitto di attribuzione di competenze sul tema oggi affrontato, ha chiaramente indicato la via a scenari legislativi del tutto innovativi e rivoluzionari. La Lega Nord ritiene che la cultura, espressa attraverso le molteplici forme di spettacolo, debba essere elemento trainante per consolidare la conoscenza delle radici culturali, storiche ed artistiche, partendo da quelle del territorio (e noi sappiamo quanto ogni campanile italiano offrire in termini di unicità e di ricchezza ai propri cittadini), e per riaffermare l'orgoglio dell'appartenenza alla propria cultura. Ecco perché noi vorremmo che la gestione e la distribuzione dei fondi statali venissero modificate in senso federale, forti anche delle sentenze della Corte costituzionale appena citate. Se il cittadino non conosce le proprie origine storiche e culturali e non ne è orgoglioso, allo stesso modo non riterrà proficuo doverle coltivare e nemmeno saprà positivamente e costruttivamente confrontarsi con esse e con le altre. La Lega Nord sa che lo spettacolo non è solo espressione di cultura: è anche industria, artigianato, lavoro, economia. La cultura esprime sempre più una buona fetta del mercato del lavoro. Una gestione più generale del FUS certamente inciderebbe in senso positivo sulle economie locali e regionali; permetterebbe alle Regioni di programmare investimenti mirati a sostenere le maestranze, gli operatori e le imprese presenti sul territorio, riequilibrando la forbice degli investimenti, ora estremamente larga, passando da un totale accentramento ad un inizio di regionalizzazione; permetterebbe alle Regioni che vogliono essere intraprendenti di richiamare l'attenzione delle grandi produzioni internazionali e dei grandi eventi musicali e culturali in genere, sul patrimonio artistico e paesaggistico che le connota; permetterebbe l'avvio di un traino positivo anche per gli operatori del turismo su tutto il territorio nazionale. La Lega Nord sa, infine, che lo Stato non può più essere considerato quale unico erogatore di risorse a favore di tutto il comparto dello spettacolo, semplicemente perché il fabbisogno complessivo nazionale di cultura andrà sempre più aumentando, semplicemente perché riteniamo

Il mecenatismo del privato, oltre che intima soddisfazione personale per il titolare, restituisce valore aggiunto al nome dell'impresa privata che ha creduto nel progetto culturale e lo ha finanziato. La Lega Nord vuole guardare oltre il mecenatismo; vorrebbe riconsiderare un privato realmente alla pari con le istituzioni, investito e coinvolto in partenariati fruttuosi e virtuosi. Un privato che possa essere attirato ed interessato ad investire nello spettacolo e nella cultura, anche attraverso condizioni di investimento innovative, favorevoli fiscalmente e stabili nel tempo. Partenariati, accordi, progetti tra privati ed enti locali, Regioni, Stato: questo può dare respiro ai 200.000 operatori del settore, che che oggi sono preoccupati perché in grande difficoltà; questo può dare carburante all'aspetto produttivo ed economico del settore dello spettacolo, a domino anche su tutti gli altri settori produttivi, *in primis* quello turistico. Per tutti i motivi esposti, consapevoli che, come sempre, la Lega Nord ha il coraggio di proporre idee innovative, non dimenticandosi di guardare alla concretezza, non dimenticandosi che tutto il comparto dello spettacolo va sostenuto e anche incentivato a produrre qualità appetibile a livello internazionale, voteremo a favore della nostra mozione e chiediamo a quest'Aula di fare altrettanto.

Presidente, signor Ministro, colleghe e colleghi, siamo in un momento particolare della vita culturale italiana. Non se ne voglia il signor Ministro se le mie parole raccoglieranno quell'atmosfera così amara e rattristata che abbiamo visto in questi giorni nelle tante manifestazioni, anche spontanee, di artisti, registi, attrici, attori, lavoratrici e lavoratori del mondo della cultura e dello spettacolo, che, davanti al Senato e alla Camera, e prima della conferenza stampa che annunciava la Mostra del cinema di Venezia, hanno voluto leggere un bel documento che noi facciamo nostro e che ha ricevuto circa un centinaio di adesioni e di firme da parte di significative associazioni. Emergenza cultura, è stato detto; Movimento emergenza cultura 2009: di questo stiamo parlando, signor Ministro, non di un taglio come gli altri. Certo, tutti i tagli danneggiano questo o quel settore vitale, ma in questo caso siamo dentro una tragedia nella tragedia, se è vero ciò che si legge e si scrive, e cioè che la cultura oggi è grande parte della nuova società e che, anzi, la società *post*-fordista e *post*-materiale dei beni comuni immateriali oggi ha bisogno di un sistema nervoso culturale assai più rilevante di quanto sia stato in passato; se è vero che scuola, università, saperi, cultura e spettacolo sono parte integrante della nuova identità culturale digitale, di quella stagione che le nuove generazioni già vivono come la stagione dei *cross-media*, dei *media* digitali, che hanno quindi più, non meno necessità di un orizzonte culturale capace di reggere alla prova del nuovo secolo. Ecco perché quello apportato non è un semplice taglio. E non si venga a dire, da parte di qualche commentatore, che è solo un accidente in un percorso che già è stato così caduco e negativo anche negli anni passati. Innanzitutto, anche una singola opera d'arte tagliata rappresenta - ce l'ha spiegato Goethe in una bella pagina dei suoi scritti - tutta l'arte nel suo insieme: anche solo un film programmato e tagliato e un'opera di teatro o di musica immaginata e non realizzata, oppure interrotta durante la *tournée*. Questo sta avvenendo in tutti i teatri italiani:

morale, prima ancora che politica. L'Italia all'estero - l'ha dichiarato anche lei - è nota per la grande opera lirica, i film, il teatro, la musica, la danza; se siamo importanti nel villaggio globale, lo si deve - me lo lasci dire - a questo e non a qualche altra figura meno simpatica.

la presidente Finocchiaro ha parlato con molta precisione. Vorrei dirle, signor Ministro, che non è un più 60 milioni di euro quello che tra breve, forse, il Presidente del Consiglio annuncerà, ma un meno 140 milioni di euro. *(Applausi dal Gruppo* *PD)*. Vorrei altresì ricordare a lei, Ministro, al Presidente,

e mezzo se si ha la capacità di accompagnare l'attività culturale con un grande indotto di turismo culturale, di attività produttive e distributive, di nuovi linguaggi creativi! Quando alle manifestazioni si presentano associazioni con ragazze e ragazzi di 20 e 30 anni che invocano di poter svolgere attività culturali per le quali non hanno spazio, dobbiamo essere consapevoli che stiamo distruggendo i nuovi gruppi dirigenti dell'Italia.

le vacche sono grigie, neanche di notte, e quando il tanto conclamato e a volte criticato Governo Prodi governò, per l'appunto, l'investimento in cultura (il FUS) aveva superato i 500 milioni di euro: VITA *(PD)*. Non sulla carta, nella realtà! E furono anche elargiti. Il Governo presieduto da Berlusconi con il suo Dicastero, signor Ministro,

per cento di investimento in cultura, a fronte del 3, 4, 5 per cento degli altri Paesi europei. Questo cosa è? Non è forse un taglio profondo alla stessa fisionomia del nostro Paese, che mai potrà competere nel mondo, nell'economia globale vendendo jeans e magliette, ma attraverso la produzione scientifica, artistica, la qualità, ridando valore ai suoi grandi talenti che malgrado tutto resistono e realizzano *film* con pochi soldi come «Gomorra», come «Il Divo» che sono premiati ai festival internazionali? Non sono sprechi, colleghe e colleghi, questa è una falsa diceria perché i soldi pubblici vanno a film come «Gomorra» che è diventato una *case history* in tutto il mondo. Gli sprechi si eliminino in altri settori! Sa, per esempio, signor Ministro - lo può dire al suo collega competente

Si, ci sono anche produzioni che piacciono a voi, colleghi della Lega. Per concludere, questo è il tema di cui stiamo parlando: investire nelle culture (meglio il plurale) vuol dire investire nel futuro dell'Italia, nella sua identità

alla morte in diretta della cultura italiana. Facciamo qualcosa per evitarla! Signor Presidente, dopo l'applauso al comiziante che mi ha preceduto,

la numerosa e nutrita presentazione di ben cinque mozioni da parte dei Gruppi politici sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), non è che un aspetto di quella crisi internazionale più ampia, che investe da qualche anno anche il nostro Paese e della quale purtroppo non si vede ancora vicina la soluzione. Sulle analisi siamo tutti d'accordo. Il settore dello spettacolo, come sappiamo, accanto al calo delle attività cinematografiche, delle produzioni teatrali e musicali, sta attraversando una fase delicatissima di evoluzione normativa e finanziaria.

quello che si sta verificando nel calcio: i più forti economicamente guidano e sorreggono il mercato, pur tra innumerevoli difficoltà (si pensi alle fondazioni lirico-sinfoniche, ai teatri stabili e alle altre grandi istituzioni culturali pubbliche e private). I più deboli, invece, sotto l'aspetto economico-finanziario (che poi non significa affatto deboli dal punto di vista qualitativo), sopravvivono invece con ancora maggiori difficoltà, acuite dall'incredibile vicenda normativa che ha in particolar modo investito il settore dello spettacolo, decentralizzando e polverizzando i finanziamenti. Se è vero, perciò, che la cultura non è un costo, ma un valore aggiunto, occorre avviare un confronto serio per fare della crisi un'opportunità di ammodernamento, un'occasione propizia di innovazione e cambiamento in cui tutti siamo chiamati a fare la propria parte. Le proteste di questi giorni portate in piazza dai lavoratori del mondo dello spettacolo sono quanto mai legittime. C'è stata una consistente riduzione del FUS che sicuramente andrà a colpire e si ripercuoterà su tutti i settori produttivi dell'arte e dello spettacolo. E, se non s'interviene per tempo, essa potrebbe avere riflessi devastanti sull'intera industria culturale nazionale. In questo senso, escludere il mondo dello spettacolo dalle misure straordinarie e temporanee di sostegno all'economia, sia pure correttamente e prontamente previste dall'Esecutivo, potrebbe essere estremamente imprudente e rischioso. Occorre invece, immediatamente, trovare in seno alle forze politiche un punto di sintesi e di convergenza tra comprensibili esigenze di bilancio e necessario sostentamento e finanziamento di un settore che rischia il tracollo. Ma in che modo intervenire? Intraprendendo con decisione la strada della valorizzazione e della crescita delle attività dello spettacolo, parte essenziale dell'identità nazionale. Il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito, com'è noto, nel 1985, è lo strumento finanziario attraverso il quale lo Stato sostiene le attività del settore spettacolo, sia del cinema sia dal vivo. Ogni anno, tale Fondo è finanziato con la legge finanziaria e viene ripartito tra i vari settori con un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. La gestione del FUS consente, inoltre, di assegnare contributi ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché di promuovere e sostenere manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero. Il FUS viene rifinanziato ogni anno con la legge finanziaria e per quest'anno il finanziamento è stato di circa 398 milioni euro. Ricordo che la dotazione per il 2007 era pari a 444 milioni. L'incerta e precaria situazione finanziaria, che interessa, in particolare, lo spettacolo dal vivo, mette a rischio la possibilità di portare a termine la riforma del settore, attesa ormai da decenni ed attualmente in discussione presso la VII Commissione permanente della Camera dei deputati. Occorre intervenire simultaneamente in entrambe le direzioni: sia, cioè, per colmare i vuoti normativi ed armonizzare il panorama legislativo stratificatosi negli ultimi decenni, sia a livello di finanziamento, onde evitare il blocco di ogni attività del settore. Lo spettacolo va considerato un'opportunità e una risorsa per l'economia, per la coesione sociale e l'immagine del nostro Paese. Insomma un valore aggiunto di una identità, di una storia e di una tradizione nazionale da valorizzare in un contesto sempre più globalizzato, indistinto, uniforme. Il settore dello spettacolo in Italia, nel suo complesso, conta all'incirca 250.000 addetti, tra artisti, tecnici, operatori, maestranze. Un'esiguità di finanziamenti pubblici, pertanto, metterebbe a serio rischio i livelli occupazionali dell'intero comparto, nonché il sistema dei diritti e degli ammortizzatori sociali. Il vuoto normativo, dunque, pesa molto. Se si vuole perciò davvero incentivare l'afflusso di capitali privati, si cominci a mettere mano a questa riforma, che tutti sollecitiamo da decenni inutilmente e che è tanto più necessaria ora, anche per fare finalmente e definitivamente chiarezza sulla divisione di competenze tra Stato ed enti territoriali. Occorre allora - come dicevo - trovare immediatamente in seno alle forze politiche un punto di sintesi e di convergenza tra comprensibili esigenze di bilancio e necessario sostentamento e finanziamento di un settore che rischia il tracollo. È questo il punto di mediazione più avanzato che si può raggiungere in un momento così difficile. Il che significa che, mentre intendiamo sostenere il FUS, dobbiamo, al tempo stesso, essere altrettanto determinati a procedere in direzione della riforma del settore. Fondamentali, risolutive e decisamente determinanti sono, allora, in questo senso, le proposte avanzate dal ministro dei beni culturali, onorevole Bondi; prima fra tutte, la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché una politica di defiscalizzazione in ambito culturale. Se questa è la direzione che auspichiamo e verso la quale intendiamo muoverci, appare del tutto evidente come l'obiettivo immediato non possa essere che quello di vincolare il Governo a rispettare l'impegno preso dai suoi componenti davanti al Capo dello Stato, disponendo con la massima urgenza uno stanziamento straordinario integrativo del Fondo unico dello spettacolo per il corrente esercizio finanziario. Pertanto, signor Presidente,

Prima di passare alla votazione delle mozioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri mattina, ha proceduto alla ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure anticrisi. È stato inoltre approvato il calendario per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Le Commissioni potranno convocarsi a partire da martedì 8 settembre. L'Assemblea tornerà a riunirsi mercoledì 16 settembre, alle ore 17, e nella seduta antimeridiana di giovedì 17 settembre per l'esame dei disegni di legge concernenti: prevenzione frodi credito al consumo; campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto; etichettatura prodotti alimentari; nonché ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione. Nella seduta pomeridiana di giovedì 17 settembre avrà luogo il sindacato ispettivo. Nel corso di tale settimana sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per la calendarizzazione delle mozioni sul Fondo aree sottoutilizzate nella settimana successiva. Le Commissioni affari esteri e difesa sono autorizzate a convocarsi, anche durante la sospensione dei lavori, in relazione a eventuali sviluppi della situazione internazionale.

approda all'Aula del Senato. L'originario testo predisposto dal Governo prevedeva un impatto sostanzialmente neutrale sul bilancio: la combinazione di entrate e uscite dava zero in termini

Le innovazioni apportate alla Camera hanno comportato addirittura un miglioramento in termini di disavanzo pari a 7 milioni di euro Il testo licenziato dalla Camera non è stato modificato da questo ramo del Parlamento nel corso dell'esame svolto dalle Commissioni 5a e 6a riunite in sede referente, né nell'ammontare, né nella composizione di risorse ed impieghi. Gli emendamenti presentati ed ammissibili sono stati respinti all'esame delle Commissioni bilancio e finanze. Rimandando alla documentazione predisposta dagli Uffici la disamina analitica dei profili finanziari del provvedimento, sono stati ribaditi quindi gli oltre 17 miliardi di euro di risorse, diversamente assicurate nel periodo 2009-2012. Da un lato vi sono gli introiti, complessivamente quantificati in 10,6 miliardi di euro, derivanti principalmente dalle misure in materia fiscale conseguenti alle intese in sede OCSE sul contrasto ai paradisi fiscali ed agli arbitraggi internazionali - che valgono circa 3 miliardi di euro a partire dal 2010 che insieme allo scudo ed altre norme di compensazione dei crediti e di ulteriore contrasto a evasione, elusione e frodi compongono un pacchetto che vale oltre 6,6 miliardi. Va qui segnalato, necessariamente, che il provvedimento reca norme per il potenziamento delle attività di accertamento e riscossione. importanti disposizioni vanno dalla semplificazione della disciplina riguardante la verifica reddituale per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 13 della legge n. 412 del 1991, alla possibilità dell'amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sui redditi e sull'IVA, di richiedere notizie, informazioni, documenti e dati di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa ad autorità ed enti che svolgono attività di controllo e vigilanza. Sono state adottate una serie di norme in ossequio alla volontà di garantire risorse senza aggravare ulteriormente la pressione fiscale, lontane dalla logica vessatoria e poliziesca nel rapporto cittadino-fisco. la norma sintetizzata come regolarizzazione delle badanti, quantificata in 1,5 miliardi di euro, norma certamente di portata più ampia, che stabilisce, infatti, una procedura straordinaria di regolarizzazione di lavoratori italiani e stranieri occupati in modo non regolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico. mediante una dichiarazione di emersione presentata da parte del datore di lavoro, previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Si tratta di una disposizione che riveste grande rilevanza per le famiglie, perché associata all'incremento del finanziamento dello Stato in favore del Servizio sanitario nazionale, nella misura di 67 milioni per il 2009 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2010, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati in base alla procedura in esame. Dall'altro lato vi sono i significativi risparmi, complessivamente quantificati in 6,4 miliardi e composti principalmente dai 2,4 miliardi della spesa farmaceutica. Le relative norme, infatti, differiscono al 15 ottobre prossimo il termine per la stipulazione della nuova intesa sulla spesa sanitaria tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e prevedono, poi, la riduzione del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale, al fine di conseguire un risparmio di 800 milioni di euro annui, che verranno destinati (mediante un fondo di nuova istituzione) ad interventi relativi al settore sanitario. di circa un miliardo per via dell'adeguamento dell'età pensionabile delle donne nella pubblica amministrazione: un primo segnale dei notevoli risparmi attesi da una misura necessaria, non solo perché adegua l'Italia ad una decisione della Corte di giustizia europea, ma perché ci costringerà a non nasconderci più dietro l'alibi che i servizi per le donne lavoratrici non ci sono in cambio di quell'ipotetico risarcimento che oramai non è più nemmeno tale. Le risorse così ottenute vanno ad alimentare diversi utilizzi, previsti complessivamente in poco più di 16,5 miliardi, concentrati nel biennio 2009-2010, con qualche anticipazione a quest'anno. utilizzi si riferiscono a misure di diversa natura: incentivi al lavoro e alle imprese, che comprendono misure per il potenziamento degli ammortizzatori sociali e l'occupazione, interventi importanti e nuovi, lontani da una logica meramente assistenzialistica perché finalizzati a mantenere in attività i lavoratori e riqualificarli affiancati da misure più tradizionali. In particolare, i soggetti titolari di trattamenti di sostegno al reddito e in costanza di rapporto di lavoro potranno essere chiamati dalle aziende di appartenenza in progetti di formazione e riqualificazione, percependo la differenza tra il trattamento e la retribuzione.

delle proroghe fino a 24 mesi della cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività; nonché, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l'incremento del 20 per cento della quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell'orario di lavoro nei contratti di solidarietà "difensivi". In tale biennio poi è prevista la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria e straordinaria, o di ammortizzatori sociali in deroga, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività autonoma o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. quindi le possibili destinazioni, nell'ambito del settore degli ammortizzatori sociali, di alcune risorse già stanziate in materia per il 2009. Al sostegno delle imprese sono poi finalizzate le disposizioni relative alla cosiddetta Tremonti-*ter*, ovvero le agevolazioni fiscali per circa 4,54 miliardi in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti in macchinari ed apparecchiature fino al 30 giugno 2010, vincolate alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali; nonché la previsione di un regime fiscale agevolato per la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone, che consente di escludere dall'imposizione fiscale, per cinque anni, il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale sino a 500.000 euro. Ulteriori interventi in favore delle imprese sono dovuti all'accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa, ma, soprattutto, dalle norme contro i ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione, una questione molto rilevante per l'intero sistema produttivo. Disposizioni in linea con quelle comunitarie, volte ad evitare in futuro eccessivi ritardi nella liquidazione di quanto dovuto per somministrazioni, forniture ed appalti, creando difficoltà di liquidità ed oneri finanziari per le imprese. Al riguardo, solo per memoria, si ricorda che nel provvedimento di assestamento del bilancio 2009, recentemente approvato, sono state a tal fine autorizzate integrazioni di cassa per oltre 18 miliardi di euro. Accanto a tali disposizioni intendo ricordare che il decreto-legge prevede ulteriori norme, a contenuto non oneroso, che rivestono un'importanza rilevantissima per un'economia a vocazione da *export* come la nostra. Mi riferisco al ruolo che potrà svolgere un nuovo sistema integrato di finanziamento e di assicurazione - la cosiddetta Export Banca - svolto con l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti e finalizzato ad abbassare il costo del finanziamento per le imprese esportatrici sulle operazioni garantire dalla SACE Disposizioni per il sistema creditizio sono contenute, invece, nell'articolo 7, che reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari, con esclusione dei crediti assistiti da garanzia o da misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici o da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato. Interventi in favore delle imprese, ed indirettamente delle famiglie, sono quelli volti al contenimento dei costi dell'energia, derivante in particolare dalla promozione dell'efficienza e della concorrenza nel mercato del gas naturale. La riduzione deriva da un meccanismo che consente una offerta a condizioni più vantaggiose. In favore delle famiglie sono certamente le disposizioni che riguardano il contenimento delle commissioni bancarie, che prevedono, a decorrere dal 1° novembre prossimo, nuovi limiti massimi per la data di valuta e la data di disponibilità economica per il beneficiario di bonifici, assegni circolari e assegni bancari, termini ulteriormente razionalizzati a partire dall'aprile 2010. A queste si accompagnano l'ammontare del cosiddetto corrispettivo onnicomprensivo vige il divieto della commissione sul massimo scoperto - pari allo 0,5 per cento e la surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta. Tra gli interventi in favore delle famiglie è, ancora, importante segnalare la spesa di 230 milioni di euro nel 2010, relativa al rimborso dei titoli obbligazionari di Alitalia, per un ammontare pari al 70,97 per cento del valore nominale, nonché dei titoli azionari sostituibili con titoli di Stato di nuova emissione, per un controvalore pari al prezzo medio nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 interventi riguardanti le pubbliche amministrazioni, e nello specifico il Patto di stabilità interno, sono previste una serie di deroghe per Regioni ed enti locali, che impegnano oltre 2,2 miliardi: ad esempio, l'esclusione dai relativi vincoli dei pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno dagli enti locali virtuosi; l'ampliamento della possibilità di spesa per Regioni e Province autonome, escludendo i pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali; la possibilità di utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, a determinate condizioni, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio. Un altro importante filone di utilizzo è costituito dalla proroga delle missioni di pace in cui sono impegnate le nostre Forze armate, per un importo di circa 510 milioni di euro, che questo decreto-legge affronta nella sua copertura finanziaria. Nell'ambito della spesa in conto capitale, va segnalato l'utilizzo di circa 209 milioni di euro per i complessivi interventi di ricostruzione a seguito del sisma che ha colpito l'Abruzzo. Si ricorda infine che le ulteriori risorse liberate dal provvedimento vanno ad alimentare il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) nel seguente modo: complessivi 11,6 miliardi per il periodo 2009-2012 e complessivi 7,7 miliardi per il periodo 2013-2017, anno dal quale decorre 1,7 miliardi. Tali incrementi, attuati mediante le maggiori risorse liberate dal provvedimento e non utilizzate, sono destinati, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013 recentemente approvato, all'attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti. *(Applausi

il decreto-legge in esame, così come ha detto la relatrice Bonfrisco, interessa una serie di misure dirette a contrastare la crisi economica in atto, nonché disposizioni per la proroga dei termini in scadenza e per assicurare la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo. sviluppo. Il provvedimento, che interviene in diversi ambiti, è stato ampliato nei suoi contenuti nel corso del passaggio presso la Camera dei deputati; quindi, sono molte le disposizioni che investono direttamente le competenze della Commissione finanze. anzitutto all'articolo 2, recante misure per il contenimento del costo delle commissioni bancarie. Tra le altre, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni bancari e circolari non può superare rispettivamente uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento; inoltre, l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non può superare lo 0,5 per cento, trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. L'articolo 4-*sexies* assoggetta all'IVA con aliquota del 10 per cento anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti il trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio. L'articolo 5 reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale, nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese, escludendo dalla imposizione il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature effettuati tra il primo luglio 2009 e il 30 giugno 2010, inclusi nella divisione 28 della tabella ATECO. È stato altresì introdotto un regime fiscale agevolato per favorire la capitalizzazione delle società, dando la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale fino a 500.000 euro per cinque anni. A tal proposito, vorrei fare alcune considerazioni sulle esigenze delle imprese e soprattutto dei cittadini del Sud, che debbono ritornare ad essere al centro dell'azione di governo. Il dibattito di questi giorni sulla questione meridionale, al di là delle opinioni personali, ha comunque raggiunto l'obiettivo di far riflettere il Governo e proporre soluzioni che vanno incontro alle esigenze di questa vasta area del Paese. un percorso nuovo che mette in campo nuovi strumenti e nuove risorse. Occorre però essere chiari su un punto: non ci dovranno più essere misure misure a pioggia, indiscriminate e sostanzialmente inutili dal punto di vista economico, ma occorrerà selezionare le infrastrutture da realizzare e le agevolazioni più efficaci. In via di esempio, per il futuro sarebbe opportuno incrementare le agevolazioni fiscali per i nuovi investimenti in impianti e macchinari, che opportunamente il Governo ha introdotto con il presente decreto-legge, misura che va sotto il nome di "Tremonti-*ter*", per gli investimenti effettuati dalle imprese del Sud. Così come occorre finalmente rinnovare il sistema bancario e finanziario con la costituzione della oggi annunciata Banca del Mezzogiorno. Si ricostruirebbe così un nuovo rapporto fra credito e conoscenza del territorio e delle imprese che nel Mezzogiorno d'Italia, andando avanti nel tempo, si è completamente dissolto,

- un suggerimento che mi permetto di indirizzare al presidente Berlusconi ed al Governo - la questione della fiscalità di vantaggio anche con meccanismi automatici di credito di imposta: si tratta cioè di scommettere sulle imprese sane e produttive del Sud, garantendo ad esse per un periodo certo e per interventi certi, incentivi concessi a fronte di iniziative serie, sostenibili, profittevoli e redditizie. Altro fattore da non sottovalutare riguarda le politiche del lavoro. Bisognerebbe offrire, in quelle Regioni che soffrono una atavica disoccupazione, la possibilità agli imprenditori di ridare opportunità lavorative ai giovani, proponendo la detassazione da tre a cinque anni dei redditi da lavoro dipendente o un'individuazione di strumenti che vadano nella direzione dell'alleggerimento del costo del lavoro. del lavoro. L'agenda dei nuovi interventi non è difficile: bisogna combattere la criminalità organizzata, sconfiggere la mala pianta dell'illegalità diffusa e puntare sulle imprese sane e soprattutto sui settori dell'agroalimentare, del turismo, delle nuove fonti energetiche, del federalismo fiscale e della ricostruzione del *welfare*. Tali azioni vanno supportate da una classe dirigente meridionale moderna ed innovativa, che abbandoni il vecchio assistenzialismo becero ed inconcludente e riporti il Mezzogiorno, anche attraverso un rinnovato regionalismo, al centro delle politiche economiche di questo e dei futuri Governi. L'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili. L'articolo 7 reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari. L'articolo 8 individua un nuovo sistema integrato di finanziamento ed assicurazione - denominato Export Banca - attraverso risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti, volto a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese, assistite da garanzia della SACE. L'articolo 10 interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti. Tra le altre cose sarà possibile, con decorrenza 2010 e tenendo conto ovviamente delle esigenze di bilancio, l'aumento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo di credito compensabile nell'anno da ciascun contribuente. L'articolo 11 prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e del Ministero del lavoro, nonché dei soggetti ad essi collegati per analisi e studi mirati all'elaborazione delle politiche economiche e sociali. reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti paradisi fiscali ed in particolare dispone che gli investimenti in attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumano costituiti - ai fini fiscali e salva la prova contraria - mediante redditi sottratti a tassazione. L'articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento ad una verifica di effettività sostanziale. introduce una disciplina (il cosiddetto scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, mediante la procedura del rimpatrio ovvero della regolarizzazione. La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera. L'operazione si perfeziona con il pagamento dell'imposta straordinaria, istituita dalla norma in esame, che consiste in un'aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere. L'articolo 14 prevede un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale, con l'aliquota del 6 per cento entro l'importo massimo di trecento milioni di euro. L'articolo 15 reca diverse disposizioni in materia di accertamento e di riscossione. Tra le altre, si semplifica la disciplina delle verifiche reddituali per determinare le prestazioni previdenziali ed assistenziali; si amplia l'ambito del pagamento rateizzato. I commi successivi, tutti aggiunti dalla Camera, dettano disposizioni varie: tra le altre, viene ampliata la base informativa di cui dispone l'Amministrazione finanziaria in sede di richiesta di misure cautelari; si concede un credito di imposta alle imprese di autotrasporto; si obbliga il PRA a segnalare all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e alla Regione i casi in cui una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli; si disciplina lo scambio reciproco di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS; si consente di affidare l'accertamento ed i controlli in materia di PREU alla SIAE; si disciplina una nuova modalità di estinzione dei debiti iscritti a ruolo di uso facoltativo per i Comuni. interviene in materia di giochi, stabilendo, tra l'altro, che il nulla osta, rilasciato dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, non collegati alla rete telematica.

L'articolo 17, tra le altre disposizioni, autorizza le Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, in presenza di eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, e proroga al 31 dicembre 2009 il periodo di tirocinio previsto per il personale delle Agenzie fiscali. L'articolo 18 prevede l'adozione di decreti del Ministro dell'economia volti a disciplinare la gestione delle disponibilità finanziarie delle società non quotate totalmente possedute dallo Stato. L'articolo 21 interviene in tema di rilascio di concessioni di giochi, stabilendo che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato debba avviare entro il 31 luglio 2009 le procedure per l'aggiudicazione della concessione agli operatori di gioco, individuati in numero non superiore a quattro, in possesso di idonei requisiti mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. L'articolo 23, tra le altre disposizioni, differisce al 30 giugno 2010 il termine previsto per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute da parte dell'Agenzia ex Sviluppo Italia; proroga al 31 dicembre 2009 il termine entro cui è consentito ai soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007 prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale tipo di servizio senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti; estende all'esercizio finanziario 2010 la disciplina sperimentale inerente i limiti di contenuto della legge finanziaria e del bilancio, introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008 per il solo 2009; modifica le modalità di pagamento dell'imposta di bollo delle cambiali. L'articolo 25 autorizza una spesa di 284 milioni di euro per la partecipazione dell'Italia a banche e fondi internazionali; interviene in materia di recupero dei versamenti fiscali e contributivi sospesi per il terremoto in Abruzzo; incrementa le risorse finanziarie destinate agli interventi di ricostruzione in Abruzzo e dispone in merito alla restituzione dei versamenti sospesi a seguito degli eventi sismici di Marche ed Umbria e di Campobasso e Foggia.

con la consapevolezza, perlomeno da parte del PD, che è stato presente massicciamente a tutta l'attività delle Commissioni, di partecipare ad una rappresentazione la la cui soluzione finale era comunque già scritta, e non era scritta in quest'Aula. Ne abbiamo avuto conferma qualche ora dopo quando, aprendo i giornali di questa mattina, abbiamo letto della decisione di porre la fiducia, comunicata evidentemente alla stampa, e di procedere immediatamente con un altro decreto. Credo ci siano problemi di forma e di sostanza, che in questo caso coincidono, per cui mi permetto di rivolgermi alla Presidenza nella sua interezza per chiedere che vengano ripristinati dei rapporti corretti, sia sotto il profilo della forma sia sotto il profilo della sostanza. Non è una semplice questione di principio; è un problema di rispetto reciproco, come in una famiglia ci deve essere rispetto tra genitori e figli e tra figli e genitori, oppure le istituzioni, da quelle familiari a quelle quale la nostra, non reggono perché scricchiolano nei fondamenti. Noi comunque, con la consapevolezza di cui ho detto, siamo rimasti a discutere per questioni di forma e di sostanza all'interno delle Commissioni bilancio e finanze.

assolutamente consapevoli. Vero è che rispetto all'impostazione di questo - credo settimo o ottavo - decreto anticrisi, le proposte che abbiamo fatto partono

tutte fondate su questo presupposto. Noi, invece, abbiamo il fondato convincimento che questo sia un altissimo rischio e che, quindi, le politiche impostate come politiche di risposta ad una crisi di breve periodo rischino di non essere assolutamente sufficienti nel caso, che si sta prospettando, di una crisi più lunga. Non amiamo iscriverci al partito delle Cassandre e men che meno essere identificati

che spero attiri l'attenzione del Governo rispetto agli assunti con cui noi affrontiamo il problema della crisi e formuliamo le nostre proposte. La crisi non sarà breve, e in questo senso nei giorni scorsi è emerso un dato significativo. Pochi giorni fa la Deutsche Bank è crollata in Borsa dopo avere annunciato che nell'ultima trimestrale aveva conseguito utili

Il crollo registrato in Borsa, altissimo, è dovuto al fatto che contestualmente la banca ha annunciato che tutti gli utili in più li metteva a riserva, perché aveva un tasso di sofferenza di mancati ritorni di prestiti alle imprese che giustificava un provvedimento di questa natura, che ha poi provocato il crollo di cui ho parlato. Che il sistema bancario lì è più scricchiolante, e quindi lo si annuncia prima, ma le sofferenze sono note anche nel nostro - cominci a fare accantonamenti nell'assunto che le imprese non riescono a ritornare dei debiti che hanno nei confronti delle banche significa che c'è un sensore molto reale, non di parte ma oggettivo e di mercato, che ci annuncia che la crisi sarà più lunga del previsto. Per questo motivo noi riteniamo che questo provvedimento contenga, sì,

caso occorre una visione più strutturale, più di sistema, in particolare per quanto concerne gli strumenti che devono essere posti in essere a sostegno del nostro sistema produttivo, perché non conveniamo sull'assunto del Ministro. La crisi non sarà breve e questi sono provvedimenti adatti per una crisi breve, per cui siamo preoccupati per la tenuta del nostro sistema produttivo di fronte a questa ipotesi. quanto riguarda le disposizioni normative riferite alle imprese, certamente la proposta di rafforzare la patrimonializzazione, e quindi gli stimoli per il rafforzamento della patrimonializzazione

ottiene dei risultati diversi, avrebbe comportato almeno due fondamentali impegni aggiuntivi: in primo luogo quello relativo alla questione dei tardati pagamenti della pubblica amministrazione, questione che riportiamo non perché amiamo ripetere come un mantra mantra alcuni concetti già sviluppati in altre sedi, ma perché oggettivamente il ritardato pagamento della pubblica amministrazione è da tutti riconosciuto, e dal Governo medesimo, come un problema che innanzitutto riguarda il ripristino della credibilità dello Stato nei confronti del sistema delle imprese.

Ancora più, rispetto a questo, resta il problema che in questa fase critica per molte piccole e medie imprese un ritardato pagamento significa un rischio mortale

quanto contenuto in queste disposizioni normative sia del tutto insufficiente ad affrontare il problema? Invito ogni collega che abbia buona volontà - lo voterà, quindi potrebbe anche leggerlo esaminare l'articolo che parla di tempestivi pagamenti alla pubblica amministrazione. La semplice lettura dell'articolo dimostra che essi non potranno essere tempestivi. Anche a un neofita della pubblica amministrazione capiterà di vedere che le procedure che si incardinano per evitare in futuro tardati pagamenti sono il presupposto per renderli più lenti.

sanzioni amministrative del tutto improbabili in una simile situazione, poiché porterebbero sicuramente alla paralisi degli atti deliberativi da parte dei funzionari. Ancora meno - vi prego di credermi - ci si può affidare alle ennesime relazioni. Credo che il Ministro per la semplificazione potrebbe opporsi a qualunque richiesta di inserire, come avviene in questo caso, in atti normativi la richiesta di pletoriche

Altra questione per noi determinante, per quanto concerne il supporto al sistema produttivo, è l'impegno del Governo a promuovere nelle sedi internazionali dovute le modifiche a Basilea 2. 2. È a tutti evidente che Basilea 2 ha un effetto prociclico; ciò, in un momento di crisi qual è l'attuale, ha un effetto deleterio rispetto alla concessione del credito.

Siccome è chiaro a tutti che Basilea 2 fonda l'erogazione del credito delle banche sulla base dei bilanci che le aziende presentano, definendo dei *rating* molto precisi, se nel 2009, sulla base dei bilanci del 2008, le aziende hanno avuto difficoltà ad avere credito, potrete facilmente immaginare che cosa capiterà nel 2010, ossia tra pochi mesi, quando presenteranno i bilanci del 2009. I bilanci del 2009 delle aziende italiane, soprattutto delle piccole e medie aziende, sono tutti al di fuori dei *rating* dettati da Basilea 2. Questa è questione cruciale per il sistema delle imprese,

anche all'interno del provvedimento in esame, come vediamo richiamate altre questioni che potrebbero non essere disciplinate dalla norma, quale l'accordo con l'ABI per la moratoria dei crediti, che credo il Governo abbia voluto inserire come forte segnale di attenzione alla questione. E veniamo a due altri aspetti su cui i nostri emendamenti si sono soffermati perché riteniamo siano questioni cruciali, non tanto

a tutti i quesiti che sono stati posti in materia, ribadendo ciò che ci si aspettava ribadisse; al momento che aveva inserito questa disposizione, ha ribadito i presupposti in base ai quali la misura la misura della tassazione della plusvalenza virtuale maturata dall'oro della Banca d'Italia doveva essere introdotta e aveva le premesse per essere perseguita.

gli italiani, nei confronti dell'oro della Banca d'Italia, credo abbiano, più o meno, lo stesso atteggiamento che gli inglesi hanno nei confronti del tesoro della Corona. Credo che al tesoro della Corona non capiti niente se viene sottratto un grosso rubino per fare cassa. Non capita niente, ma non si fa.

grandi capacità nella gestione del bilancio e nel reperire le risorse necessarie, pure in un momento di difficoltà, voglio credere che non gli mancassero altri modi per trovare 300 milioni di euro.

la Corte dei conti è un'istituzione di garanzia. Tuttavia, credo che moltissimi amministratori con cattive intenzioni - purtroppo, ve ne sono - siano più intimoriti dalla magistratura contabile che dalla magistratura ordinaria. Credo che la Corte dei conti sia un'istituzione che ad oggi ha prestigio e capacità di intervento. Legare in questo modo le mani alla magistratura contabile non è un bel servizio, né nei fatti, né nella forma, né nella sostanza. Per tale motivo su questo punto ieri sera abbiamo fortemente dibattuto in Commissione. Abbiamo poi appreso dai giornali - quindi, non sapendo mai se siamo nella realtà o nella rappresentazione, ciò avveniva fuori da questa sede - che c'è l'intendimento di intervenire, e non possiamo che compiacercene. Richiamo infine due aspetti.

rappresentato con molta forza il principio cardine della certezza sulle risorse: togliere di torno alla questione Abruzzo il dubbio che vi siano risorse virtuali e la sensazione sul territorio che le risorse virtuali non potranno essere messe adeguatamente a disposizione e, quindi, che gli abruzzesi potranno essere costretti ad affrontare l'inverno in condizioni assolutamente disagiate.

Come si è detto per altri punti di questo decreto, intervenire rapsodicamente sui problemi non rende un grande servizio, perché fa perdere la visione contestuale e di insieme.

gare vinte al massimo ribasso laddove è evidente che imprese sane non possono permettersi altrettanto ribasso. Forti dubbi restano quindi sull'efficacia di questo strumento per combattere problematiche di tale natura. Si tratta di un problema che richiede un approfondimento serio e una capacità globale di affrontare la questione in tutta la completezza che ho anche qui richiamato. Il *day by day,*

soffermeranno su altre problematiche. Ricordo, tra tutte, lo scudo fiscale, questione su cui c'è profonda divergenza tra il Gruppo del PD e il Governo. Concludo, signor Presidente.

Abbiamo avuto la precisa sensazione che si ritenesse di procedere diversamente, quindi con un aggravio assai oneroso, per l'impossibilità di portare alla Camera questo provvedimento la prossima settimana. Non è positiva per l'immagine che diamo all'esterno l'idea che, poiché una parte del Parlamento della Repubblica ha la valigia in mano, non si riesca a fare oggi quello che si deve fare oggi, nel punto in cui lo si deve fare.

di 3 milioni di euro, "spannometricamente" contati, e tutto questo perché non ce la siamo sentita di togliere la valigia dalle mani di chi la settimana prossima, alla Camera, una nuova finestra"). Comunico che sono state presentate quattro questioni pregiudiziali. Ha chiesto di intervenire il senatore Casson per illustrare la questione pregiudiziale QP1. *(PD)*. Signor Presidente del Senato, signori senatori, signori del Governo, mi accingo ad affrontare una questione pregiudiziale di costituzionalità del decreto-legge al nostro esame che ha del paradossale, direi che è quasi una questione dagli aspetti per certi versi kafkiani. Sappiamo tutti in Senato e soprattutto lo sapete bene voi, signori del Governo, che state proponendo l'approvazione di alcune norme sulle funzioni e sulle attività della Corte dei conti che sono palesemente viziate - sottolineo, palesemente viziate - da profili di illegittimità costituzionale. Sapete altrettanto bene di aver già predisposto, come Consiglio dei ministri, un decreto-legge correttivo di tali vizi che interverrà dopo che avrete costretto i vostri senatori a votare delle norme palesemente incostituzionali, e consapevolmente. Ciò per evitare l'inevitabile e immediata bocciatura, almeno sul punto, da parte del garante della nostra Costituzione. Lo sapete benissimo. Eppure procederete come se nulla fosse, come se delle regole, delle leggi ordinarie e della Costituzione si potesse tranquillamente fare a meno, giocando con norme e pandette come fossimo al gioco delle tre carte. A conferma di questo vostro gioco perverso, ricordo in quest'Aula il parere, l'invito rivolto ieri al Parlamento ed al Governo in Commissione giustizia dai senatori della stessa maggioranza, certamente non ciechi di fronte ai palesi vizi di legittimità costituzionale da noi segnalati *in parte qua*. I senatori di maggioranza segnalavano di valutare «la congruità rispetto al quadro costituzionale delle innovazioni alla disciplina della Corte dei conti apportate dal disegno di legge di conversione in esame (...), in particolare sotto il profilo del nuovo strumento di controllo preventivo di legittimità, del controllo nomofilattico vincolante affidato alle sezioni riunite della Corte dei conti su richiesta del primo Presidente (...), della possibile disparità di trattamento tra i funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato e quelli delle amministrazioni regionali e periferiche in ordine all'esonero da responsabilità contabile (...) e, infine, della disposizione (...) che (...) stabilisce la nullità di qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere relativamente ad atti qualificati (...), diversamente dal dolo e dalla colpa grave, col rischio di paralizzare l'azione investigativa del pubblico ministero contabile Si tratta esattamente degli stessi vizi da noi chiaramente segnalati ieri in Commissione ed oggi in sede di pregiudiziale in quest'Aula. Bisognerebbe semplicemente prenderne atto nell'interesse delle istituzioni e della giurisdizione. Purtroppo sappiamo che non sarà così. così. A parte il vostro consueto vizio di fare strame dell'articolo 77 della Costituzione, che vi fa completamente sottovalutare, se non proprio eliminare, i requisiti della necessità e dell'urgenza (cosa c'entrano ad esempio con il decreto-legge le norme sulla composizione del Consiglio superiore della magistratura militare e quelle sulla Corte dei conti non lo sa nessuno), a parte il vostro ulteriore vizio di inserire in un decreto-legge disposizioni nuove e disomogenee ad *iter* parlamentare già avviato, così comprimendo in modo irragionevole il previsto controllo del Presidente della Repubblica, nel decreto-legge al nostro esame avete altresì inserito le norme sulla Corte dei conti criticate - dicevo - da senatori della vostra stessa maggioranza ed in assenza di qualsiasi requisito di necessità, di urgenza, di omogeneità rispetto al tipo e al titolo delle norme introdotte dal presente decreto-legge. In particolare, il comma 30 dell'articolo 17, selezionando irrazionalmente gli atti e i contratti da sottoporre al controllo preventivo di legittimità Corte dei conti, crea una evidente disparità di trattamento tra lo Stato e gli altri enti, di cui all'articolo 114 della Costituzione, così violando palesemente sia l'articolo 3 che lo stesso articolo 114 della Costituzione. Inoltre, con l'introduzione del comma 30-*ter* dell'articolo 17, il procuratore contabile può esercitare l'azione contabile solo in presenza di una specifica e precisa notizia di reato, cagionato per dolo o colpa grave, e il danno all'immagine sarà perseguibile solo in caso di sentenza irrevocabile di condanna, così riducendo sensibilmente il margine di intervento delle procure contabili, se non proprio eliminando in tanti casi il controllo contabile stesso.

sancisce l'esclusione della gravità della colpa in determinate situazioni. Questa norma, assieme alle norme di carattere generale che ho indicato, crea inevitabilmente vere e proprie zone franche nell'accertamento degli illeciti e delle relative responsabilità amministrativo-contabili nella gestione delle risorse pubbliche, così violando il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione e, segnatamente, il principio di responsabilizzazione degli amministratori e dei dipendenti pubblici,

Infatti, la proposta composizione nominativa delle sezioni riunite contrasta con il principio di autonomia e di indipendenza che l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione assicura ad ogni magistrato contabile che eserciti la funzione di controllo, oltre che con un'evidente principio di razionalità e di logicità che da tempo la giurisprudenza della Consulta ha assunto ad ulteriore parametro di costituzionalità. Sempre con riferimento a questo comma 31, devo osservare che la previsione di pronunce di carattere generale (o di «orientamento», come dite), se può giustificarsi in presenza di orientamenti contrastanti tra le diverse sezioni regionali di controllo, non si giustifica certamente in mancanza di contrasto. Questa previsione normativa espropria di fatto - espropria, lo sottolineo - le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti delle proprie competenze legislativamente determinate su base territoriale, attraendole a livello centrale proprio nei casi, peraltro del tutto indeterminati, ritenuti di maggior rilievo o delicatezza, pur in assenza di ogni contrasto o incertezza interpretativa. Tale previsione si pone altresì in controtendenza con i principi desumibili dal già richiamato articolo 114 della Costituzione, da cui discende, tra l'altro, l'articolazione della funzione di controllo esterno a livello regionale e locale. Inoltre, la funzione di orientamento generale renderebbe anche superflua ogni successiva pronunzia delle sezioni regionali, svuotandole di fatto di funzioni significative. E sul punto sarebbe proprio interessante sapere che cosa ha da dire il partito della Lega Nord. Segnalo, infine, che il presente decreto‑legge prosegue nel tentativo - a nostro modo di vedere perverso - di gerarchizzazione della Corte dei conti già parzialmente realizzato, e da noi contestato, con la legge 4 marzo 2009, n. 15 (la cosiddetta legge Brunetta), che ha modificato la coerenza del sistema costituzionale di controllo esterno della Corte dei conti, controllo che viene ora ad essere asservito e subordinato ai Governi centrali e locali, a detrimento del corretto rapporto con le Assemblee parlamentari e con le assemblee elettive territoriali. Il presente decreto‑legge, pertanto, così come ha già fatto la legge n. 15 del 2009, interviene di nuovo pesantemente sulle funzioni e sull'ordinamento della Corte, in contrasto con le esigenze e con le garanzie poste dalla Costituzione, nonché con i principi posti a presidio delle magistrature, continuando a introdurre principi e criteri gerarchici e accentratori in modo non compatibile con i richiamati principi costituzionali. Pertanto chiediamo che, preso atto di tali evidenti e palesi profili di illegittimità costituzionale, il Senato deliberi, ai sensi dell'articolo 93 del proprio Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1724.

finestra") *(PD)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi del Senato, signori del Governo, il decreto-legge di cui oggi si discute la conversione in legge contiene norme di notevole rilevanza economica in funzione anticrisi e dispone all'articolo 1-*ter* una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri occupati irregolarmente nell'attività di assistenza di componenti della famiglia cito testualmente - «affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza» o che svolgono «lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare». La regolarizzazione avviene mediante una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Rispetto a questa norma, il Gruppo del PD solleva una questione pregiudiziale, rilevando la manifesta violazione del principio di uguaglianza sancito dell'articolo 3 della Costituzione, per ragioni assai evidenti e che tra un momento illustrerò. Prima di farlo vorrei però avanzare alcune considerazioni generali. La prima riguarda la materia trattata - cioè l'immigrazione e la condizione di irregolarità - e l'invito all'emersione dei lavoratori stranieri che si trovano in condizione irregolare. il Governo ammette implicitamente la rilevanza del lavoro immigrato, del quale proprio non si può fare a meno, tanto che occorre far violenza alla legge e alla normativa, perfino a quella approvata solo da qualche settimana, e fresca d'inchiostro, contenuta nel cosiddetto pacchetto sicurezza. Con quel provvedimento - è bene ricordarlo a chiare lettere - oltre ad inserire nel nostro ordinamento una normativa inapplicabile nella pratica (e questo è il male minore, al quale abbiamo ormai un secolare allenamento), si è voluto affermare un principio che fa fare parecchi passi indietro alla nostra civiltà: chi entra in Italia, o viene a trovarsi sul territorio nazionale, senza i regolari documenti compie un reato. Si è dunque criminalizzata una situazione che è quasi sempre il risultato della necessità, e spesso la conseguenza della farraginosità della nostra legislazione in ambito migratorio. Ci auguriamo, a questo proposito, che l'Italia, "Patria del diritto", come dice la retorica, possa disconoscere presto la paternità di questa norma e di altre norme incivili, come l'aggravante di pena per gli irregolari, mediante l'intervento della nostra Alta Corte. Ma adesso il Governo fa una clamorosa inversione a U: non solo regolarizza il rientro di capitali illegalmente esportati con l'obolo dell'1 per cento sul valore, ma regolarizza anche chi è entrato (non uscito) illegalmente, mediante il versamento all'erario di un contributo di 500 euro. Poiché, in molti casi, l'onere del pagamento sarà traslato sulle spalle dell'immigrato (che dovrà pagare anche per il permesso di soggiorno), ricordo ai colleghi che si tratta di un importo pari ad almeno il 5 per cento del reddito annuo dell'immigrato regolarizzato. Chiediamo infatti a chi sostiene un invalido o alleva un bambino - e fa un lavoro utile ed indispensabile, come riconosce questa stessa legge - un contributo almeno quintuplo di quanto non venga chiesto al contribuente infedele che ha frodato il fisco e ingannato il suo Paese. La seconda considerazione generale è che questa sanatoria parziale e selettiva - mi spiace per gli amici della Lega, che a questa parola forse sobbalzano sullo scranno, ma di sanatoria si tratta - trova la sua giusta collocazione in un decreto anticrisi. Infatti, è proprio vero: il *welfare* familiare italiano è in grave crisi, perché i trasferimenti pubblici per famiglia e figli sono, da noi, solo una frazione di quelli operati dagli altri paesi dell'Unione europea (si consultino a questo proposito i dati di EUROSTAT, di cui posso fornire l'indirizzo *web*, se richiesto). Ora, per tutelare questa famiglia in crisi il Governo ha scelto non di riformare gli iniqui criteri di ripartizione tra le famiglie degli scarsi trasferimenti pubblici, ma di contraddire la normativa che ha trionfalmente imposto al Paese solo qualche settimana fa. Con la terza considerazione generale ricordo che questa maggioranza ancora una volta smentisce se stessa. Le norme contenute nei vari involucri del pacchetto sicurezza avevano un doppio obiettivo. Il primo era quello di rendere più tortuosa, impervia e difficile la vita dello straniero nel nostro Paese. Riconosco che questo obiettivo è stato magistralmente centrato: la missione è stata compiuta al 120 Il secondo obiettivo era la "deterrenza": un principio per lo meno discutibile, come sanno bene gli esperti e gli studiosi di queste materie, e che spesso non funziona. È certo, però, che la deterrenza funziona ancora meno quando i potenziali autori del reato si accorgono che la norma non viene attuata, o viene sospesa o, comunque, disattesa. Così, i ripetuti condoni in materia impositiva, fiscale o edilizia hanno nutrito l'italica schiera di esportatori di capitali, evasori fiscali e costruttori senza scrupoli. Non sarà così anche per le famiglie, intrappolate tra le necessità familiari e l'impervia normativa migratoria, che rende loro difficile impiegare regolarmente il lavoro straniero?

Non ci sarà forse qualche magagna nelle politiche migratorie, riconducibile non a leggi troppo blande ma a leggi sbagliate? Torniamo all'articolo 1-*ter*, che opera una serie di irragionevoli discriminazioni. Queste riguardano sia i lavoratori stranieri interessati dalla regolarizzazione, sia i requisiti che i lavoratori stessi devono avere per essere regolarizzati, sia, infine, i datori di lavoro che possono effettuare la dichiarazione di emersione. È in queste discriminazioni (si veda il primo comma dell'articolo in questione) che risiede la manifesta violazione del principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione. La dichiarazione di emersione, infatti, non è estesa a tutti i lavoratori irregolari, ma riguarda solo quelli che svolgono attività di assistenza e di sostegno alle famiglie. Non c'è ragionevolezza in questa disposizione: l'irregolare emerso, infatti, ottiene la sospensione del procedimento penale (per ingresso clandestino), l'estinzione del reato e, quindi, il permesso di soggiorno. Ma chi è l'irregolare così beneficiato? Non qualsiasi immigrato, e nemmeno un immigrato lavoratore qualsiasi, ma - diciamo così - l'immigrato "di famiglia". La sua regolarizzazione dipende dalla professione svolta, con un criterio profondamente discriminante. Forse che il muratore irregolare, che contribuisce alla costruzione della casa nella quale abiterà una famiglia, svolge una funzione meno utile di quella della *baby sitter*, ugualmente irregolare, che accompagna il bambino di quella stessa famiglia all'asilo? Forse che l'irregolare proveniente dall'India, che munge le mucche di una fattoria padana e contribuisce a produrre il latte che berrà il bambino di quella stessa famiglia, compie una funzione socialmente meno rilevante? Lascio all'immaginazione dei colleghi il compito di formulare altri possibili esempi. Ma è questa discriminazione che determina «l'esito paradossale e senz'altro incostituzionale di far dipendere la rilevanza penale di un comportamento, e l'applicazione delle conseguenti sanzioni penali, dalla professione e dalle mansioni svolte dal lavoratore straniero». in base a questo articolo, commetterà un reato se svolge attività di cuoco, di giardiniere, di muratore o di mungitore, ma non violerà la norma penale se accompagna un bambino a scuola o una persona anziana a passeggiare. il mio tempo stia per scadere e non mi addentro in ulteriori considerazioni, peraltro contenute nel testo della questione pregiudiziale a vostra disposizione. Ma credo che la manifesta violazione dell'articolo 3 della Costituzione sia motivo più che sufficiente per indurre i molto onorevoli e ragionevoli colleghi di questo emiciclo

Ha chiesto di parlare il senatore D'Alia per illustrare la questione pregiudiziale QP4. la giornata di oggi ha un contenuto manifestamente surreale. Siamo chiamati a celebrare un rito codificato dai nostri Regolamenti e dalla Costituzione, sapendo benissimo che è solo un rito, perché

afferenti le pregiudiziali di costituzionalità che riguardano articoli di questo provvedimento che il Governo si appresta a modificare proprio per evitare

abbastanza paradossale, in cui svolgiamo il gioco delle parti avendo noi torto e voi ragione, sapendo però voi di avere torto, tant'è che ci darete ragione domani, ma dandoci torto oggi.

Sappiamo che la nostra democrazia ha due ha due presìdi fondamentali e caratterizzanti: uno è il Parlamento, l'altro è la Costituzione. Ciò che distingue le democrazie dagli altri regimi possono essere i treni che arrivano in orario, può essere un ponte costruito al punto giusto e che non cade; ma ciò che distingue alla radice le democrazie da altri sistemi è la centralità del Parlamento, il riferimento alla Carta suprema che è la nostra Costituzione. Sappiamo altresì, perché questo è nella cronaca che scriveremo di questa giornata, che poi si metterà la fiducia su questo disegno

E il Parlamento assicurerà la fiducia su un provvedimento sfiduciato dal Governo, che nel frattempo lo

È il contrario della fiducia! Non si può chiedere una fiducia su un atto sfiduciato dal Governo! Vi rendete conto del paradosso e del rito che stiamo svolgendo nel nome della democrazia? Questo non c'entra niente! Si tratta di un'alchimia costituzionale, non c'entrano la Costituzione e la democrazia. Sono alchimie, dipenderà dal numero che verrà assegnato, in sede di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, da parte del Poligrafico dello Stato.

strano giro? Se il Governo è convinto di dover modificare alcune norme che ha appena licenziato,

i profili di non costituzionalità del provvedimento comma 11, si prevede l'estinzione del reato di soggiorno irregolare nonché dei reati commessi dai datori di lavoro. In realtà, l'estinzione del reato è un'amnistia: si deve prevedere la non punibilità. Se si prevede l'estinzione, si rientra nell'ipotesi prevista dall'articolo 79 della Costituzione, cioè l'estinzione del reato è un provvedimento di amnistia e serve il voto qualificato dei due terzi dei

dovuto assolvere il compito di recare una serie di misure per alleviare la situazione economica e sociale di questo Paese in un momento di crisi internazionale e nazionale. dunque avviata la discussione in Parlamento e nelle competenti Commissioni di merito, che affrontarono questo tema e modificarono il testo del decreto.

stata posta la fiducia. Tale maxiemendamento conteneva una serie di norme che modificavano il testo approvato dalla Commissione. Il presidente della Camera Fini, in un accorato intervento di natura istituzionale, ha lamentato la difficoltà di garantire un esame parlamentare del decreto;

Fra le tante abnormità, ve ne sono alcune molto gravi che, peraltro, avrebbero dovuto scandalizzare i colleghi della Lega. Mi riferisco, in particolare, alle norme sulla Corte dei conti. Infatti, cari colleghi,

eventuali danni all'erario e quindi ai contribuenti. Tali norme, infatti, precludono alla Corte dei conti la possibilità di esercitare quel controllo giurisdizionale che la Costituzione e le leggi italiane le attribuiscono, perché questo è contenuto nel decreto. è contenuto nel decreto. Tali norme rendono inutile l'esercizio dell'azione contabile, rendono inutile l'accertamento della responsabilità amministrativa

ora cosa succede? Vi siete accorti, perché qualcuno autorevolmente lo ha fatto presente, che tutto ciò non può andare. siete stati ostinati, perché avete dimenticato che, nel promulgare il cosiddetto pacchetto sicurezza, il Capo dello Stato ha inviato una lettera al Governo nella quale ha sottolineato l'impossibilità di esercitare le sue prerogative costituzionali di fronte ad un insieme di norme eterogenee, alcune delle quali importanti ed utili al Paese, altre in aperto contrasto con la Costituzione.

di esercitare quelle funzioni, proprie di una democrazia moderna e civile, che la Costituzione loro assegna nel nostro Paese! Questo è il punto di rottura, sotto il profilo costituzionale, del decreto e dei precedenti atti che voi, a colpi di maggioranza, avete approvato. Questa è la crisi del sistema costituzionale del nostro Paese e del modo con cui si articola il rapporto tra Parlamento, Esecutivo e Capo dello Stato.

o come decreto-legge o come disegno di legge, o in sede di conversione o in sede di esame parlamentare, agganciate "vagoni" che sul piano dei contenuti non hanno alcun significato e alcuna coerenza rispetto al testo proposto. In questo modo impedite, non solo al Capo dello Stato di fare le sue valutazioni su quel testo, perché è chiaro che egli egli non può fare un rinvio parziale di una legge, ma anche ai cittadini di comprendere se realmente stiate adottando un pacchetto di norme che ha la sua efficacia ed è produttivo di effetti positivi per il Paese. Fate solo degli *spot*. *spot*. Tutto questo sul piano politico può essere censurabile, ma sul piano istituzionale e costituzionale non è più sopportabile. Non lo è perché in un sol colpo avete scardinato tutti i sistemi di funzionamento nel rapporto tra l'Esecutivo ed il Parlamento. Questo è l'elemento critico che noi abbiamo sintetizzato nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, alla quale rinvio, facendo solo un esempio: la regolarizzazione di colf e badanti. Anche questa norma, così come l'avete concepita, è ipocrita. Infatti sapete bene che l'unica operazione di emersione dal lavoro irregolare è quella contenuta in questa disposizione,

irregolari, ma solo con riferimento a questo settore di attività lavorativa, lasciando fuori gli altri lavoratori irregolari, e agganciando a questo il presupposto di fatto su cui si dovrebbe applicare una norma penale che avete introdotto, quella sull'immigrazione clandestina. Quindi, anche sotto questo profilo introducete un sistema in forza del quale il presupposto di fatto differenziato e discriminato nel determinare l'applicazione o meno di una sanzione penale. Non credo che tutto ciò meriti particolari commenti, se non quello che siete arrivati al capolinea

fra Governo e Parlamento, ma anche nel modo di interpretare in maniera assolutamente opaca e non trasparente il rapporto fra il Governo, il Parlamento e i cittadini che vi votano.

Il collega Livi Bacci ha parlato di fallimento delle politiche di governo dell'immigrazione in Italia. Su questo siamo perfettamente d'accordo.

Certo, sul tema dei controlli preventivi di legittimità ci sono forti perplessità; però ricordiamo che questo si pone all'interno di un provvedimento che ha misure antirecessive importanti ed urgenti, che quindi richiedono un'immediata conversione in legge di tale provvedimento. avremo tempo e modo, anche alla luce del decreto correttivo che a breve entrerà in vigore, di valutare complessivamente il tema. Vorrei far notare, ma senza volontà di fare polemica, che ho esaminato attentamente gli emendamenti dell'opposizione sull'articolo 17, per valutare se ci fosse una proposta alternativa alle norme del Governo in materia di responsabilità contabili, ma non ho trovato null'altro che emendamenti soppressivi. Ciò è forse non c'è una volontà reciproca di studiare il tema, di approfondirlo, di non lasciarlo più disciplinato in maniera confusa e basata su singole giurisprudenze delle sezioni regionali della Corte dei conti, ma di cercare di trovare una

*(PD)*. Signor Presidente, colleghi, credo che, se Kafka fosse con noi su questi banchi, si sentirebbe piccino e frustrato, perché neppure il suo genio, pur contorto, avrebbe mai pensato di riuscire ad inventare un tale labirinto istituzionale, un tale guazzabuglio normativo come quello che abbiamo avuto di fronte oggi e nelle ultime settimane. I colleghi Casson, D'Alia, Li Gotti e Livi Bacci hanno illustrato alcune questioni pregiudiziali. Le voteremo tutte, ma mi consentirete di insistere su un punto,

Non ho però capito se intende porre mano anche a quest'altro obbrobrio giuridico previsto: mi riferisco alla questione toccata proprio adesso dal collega Mazzatorta. Onorevole collega, signor Presidente, mi spiegherò con un esempio, così ci capiremo

e provenienti da fuori Europa, che costoro, per il solo fatto di essere nati altrove e di trovarsi a calcare il nostro territorio, sono fuorilegge. Ma quale legge hanno violato? Nessuna, a meno che abbiano commesso delitti già previsti, e loro non ne hanno commessi.

Ma la nostra penisola contiene già centinaia di migliaia di immigrati, che non hanno il permesso di soggiorno ma l'hanno chiesto lealmente da tempo intanto svolgono un lavoro. Essi hanno depositato presso le nostre questure i loro nomi e cognomi e quelli delle loro famiglie, nonché i nomi e i cognomi dei datori di lavoro, cittadini italiani, e tutte le indicazioni sui luoghi e le modalità del lavoro. Si 140.000 persone ed 80.000 sono state respinte. Le altre sono nel limbo, ma sono precipitate nell'inferno perché nel frattempo si è varato il nuovo reato di clandestinità. Ovviamente, chiamarli clandestini, in una simile condizione, è un caso tipico di quell'irresistibile impulso alla comicità e al paradosso per il quale la nostra penisola è famosa. migliaia di persone straniere di cui si sa tutto nelle questure e nelle prefetture, e che figurano spesso nei record del nostro mercato del lavoro (per esempio, in testa alle classifiche delle morti sul lavoro che, sempre per quel tipico senso dell'umorismo, chiamiamo «morti bianche» benché siano orribilmente rosse di sangue e nere di vergogna), queste persone sono anche delinquenti. Per contagio automatico tra reato dell'immigrazione irreale e reato complementare del datore di lavoro italianissimo, anche il datore di lavoro è favoreggiatore ed anche lui è fuorilegge-criminale. Allora, poiché la questione era un po' troppo grossa, si è deciso l'antidoto, grazie anche alla nostra azione, di cui andiamo fieri, perlomeno colf e badanti saranno regolarizzate: dunque, centinaia di migliaia di persone, italiani e non italiani. Nel fare questo però succede il patatrac totale. Vi faccio un esempio. I coniugi Bricolo o Mazzatorta, residenti a Varese, gestiscono un ristorante. Hanno alle loro dipendenze da tempo i coniugi Ibrahim, in nero, perché non riescono a legalizzarli: la signora Fatima Ibrahim fa la colf e la badante, e pertanto sarà regolare, e con lei metà del signor Bricolo; il marito Isham, invece, che fa il cuoco nel ristorante, è criminale, non sarà legalizzato e la metà del signor Bricolo, datore di lavoro, sarà pure criminale. Quindi, il signor Bricolo sarà a metà legale e santo, a metà fuorilegge, che non è male come condizione, salvo poi dover chiamare l'autoambulanza per aiutare il signor Bricolo a capire qual è la sua identità. Cari colleghi, voi li regolarizzerete, farete un'altra sanatoria ad ottobre perché tutto questo non è accettabile, per discriminazione dei vostri italianissimi concittadini che sono a metà criminali e a metà regolari.

i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza discriminazione di sorta, senza distinzione di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ceto, di nascita o di altra condizione. È necessario aggiungere un'altra formula? Sono tutti uguali, eccetto: idraulici, edili, pastori d'alpeggio, cuochi, barcaioli, raccoglitori stagionali di pomodori, posteggiatori, scalpellini di pietra serena, eccetera eccetera. Questo voi state dicendo. È una pazzia, una pazzia giuridica e, prima che giuridica, logica e morale, e voi volete votare questa pazzia. Mi rivolgo a voi, colleghi di questo Parlamento umiliato ed offeso: esiste ancora in noi, in voi, la memoria e l'orgoglio di ciò che anima la legge e la rende sacra, e cioè la sua dirittura, la sua chiarezza e semplicità, la sua universalità, il suo rispetto per coloro cui dovrà applicarsi e, prima ancora, per coloro cui spetta la responsabilità terribile ed emozionante di promulgare la legge? Nonostante tutto, abbiamo ancora fiducia che possa avvenire, che la coscienza parli ancora in ciascuno di noi e in noi tutti insieme, ma soprattutto in voi, colleghi della maggioranza. Voi oggi siete chiamati a votare una cosa e tra tre settimane voterete il contrario. Ma come è pensabile? Credo che il Governo abbia bisogno che per un momento voi diciate no. Siete voi che dovreste dirlo. che non si legifera con questa sciatta arroganza, che crea solo confusione nei cittadini, nei nostri e nei vostri elettori. Voi dovreste aiutare il Governo ad avere, certo, l'urgenza dei problemi, ma non la fretta dell'azzeccagarbugli. E questo non ha nulla a che vedere col buonismo, né col lassismo, né col veteroterzomondismo; ha a che vedere con la legalità come metodo di governo dei fenomeni. che ciò che era giusto sia ancora possibile; che ciò che era giusto, nobile e sensato all'origine della nostra istituzione non sia ormai, per dirla con Jonathan Swift, cancellato, né degradato nella corruzione. Questo è il senso del Parlamento, non della maggioranza o dell'opposizione. Questo è il senso delle prerogative parlamentari: saper dire al Governo, quando il troppo è troppo, che non si possono varare tre decreti a catena per salvare un primo *vulnus*. Credo che spetterebbe innanzitutto a voi dire al Governo: badate, questa è forse la strada del consenso facile, ma demagogico e controproducente.

Signor Presidente, scuseranno i dotti colleghi se a rispondere son io, che non sono certamente un giuscostituzionalista. Ma forse, anche perché i problemi di tipo costituzionale non sono ben posti, abbiamo pensato di non scomodare i nostri campioni esperti di Costituzione, anche in questo mutuando - me ne scuseranno i colleghi - quel che Churchill diceva a proposito della guerra, cioè che è una cosa troppo importante per farla fare soltanto ai generali, per cui, in questo caso, permetteranno che

l'altra concerne il sistema di copertura che, veniva eccepito, non è coerente con la legge di contabilità. In ordine a questi due problemi non avete ritenuto di dover continuare a parlare, ed è chiaro ed evidente il perché. Per quanto riguarda i sistemi di copertura e la contrarietà alla legge di contabilità, per molti dei casi citati questi erano dovuti al fatto che l'assestamento non era stato ancora votato, ed invece ieri,

quello dello scudo fiscale, probabilmente coloro che oggi hanno parlato di badanti e di Corte dei conti sanno benissimo che se aveste continuato a governare voi, se avesse continuato a governare Visco, sarebbe entrato nell'ordinamento il divieto di effettuare in contanti qualsiasi transazione di importo superiore a 100 euro. La tracciabilità sarebbe stata totale, ed era il motivo per cui tutti i capitali sono andati via, ed il motivo per cui oggi dobbiamo intervenire per far ritornare quei capitali, per dare coraggio all'intrapresa e ai risparmiatori e per continuare di nuovo ad investire, così come in due anni non si era fatto. Così come non si erano realizzati i cantieri e come oggi è difficile, come ha detto il senatore Musi, che vi siano interventi in conto capitale, perché per effettuare gli interventi in conto capitale bisognava che vi fossero i progetti: i progetti che voi, per due anni, avete dimenticato di effettuare, perché

della Corte dei conti potremmo parlare a lungo. Anzitutto, ci piace molto la difesa che ne avete fatto, trattandosi di un organo che trova le sue radici nella legge n. 100 del 1924,

nessun'altra possibilità per approvare quello che nella buona sostanza - mi riferisco alla buona sostanza tante volte invocata da voi - non è un provvedimento sulla Corte dei conti

un momento di facezie: il Popolo della Libertà ha sede in Via dell'Umiltà, ma ogni tanto un po' di presunzione lasciatecela avere! La nostra presunzione è che stiamo facendo quello che vogliono gli italiani. Per questo rigettiamo le vostre proposte di incostituzionalità, le vostre pretese di bloccare un processo di innovazione che questo Governo molto pazientemente ed abilmente sta portando avanti. Per questo voteremo no alle vostre questioni pregiudiziali.

Presidente, non credo di rendere una comunicazione inattesa. A questo punto dei lavori parlamentari, il Governo, che attribuisce grande importanza importanza a questo provvedimento, appone anche in questo ramo del Parlamento la questione di fiducia per l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa. La Conferenza dei Capigruppo, all'unanimità, ha organizzato il dibattito sulla fiducia. Procederemo quindi come segue: oggi, alle ore 16,30, avrà inizio la discussione sulla fiducia, che durerà fino alla sua conclusione. Domani, alle ore 9, dichiarazioni di voto e voto di fiducia.

lo scorso maggio all'ospedale di Aosta, dov'era ricoverato da qualche giorno. La spedizione era guidata dal geologo Ardito Desio. Penso sia importante ricordare questa impresa, ma anche i tanti alpinisti italiani morti, sia sulle nostre cime che in quelle famose di tutto il mondo, come la giovane alpinista vicentina

Cristina e Giampaolo avevano conquistato il K3 27 anni dopo che lo scalatore vicentino Renato Casarotto, morto in un crepaccio sul K2 nel 1986, era salito per primo lungo lo spigolo Nord del Broad Peak, ovvero Cima Larga, il K3. A loro va con grande affetto il nostro

Intervengo per esprimere il mio profondo disagio, che è stato veramente pesante e insopportabile, nel corso della seduta pomeridiana del 29 luglio scorso. Presidente, nel corso di quella seduta sono avvenuti due eventi, inconcepibili e di assoluta gravità per l'istituzione che rappresentiamo, senza che dalla Presidenza del Senato, né dai Gruppi, né dall'Aula ci sia stata una reazione. Il primo fatto nel corso dell'intervento della collega Bugnano, che rilevava semplicemente l'assenza del ministro Bondi, il sottosegretario Giro ha avuto un comportamento scomposto e offensivo nei confronti del Senato della Repubblica. Il secondo fatto, conseguenza del primo, è che, mentre il senatore Russo richiamava con una certa foga il Sottosegretario ad un atteggiamento più rispettoso, il senatore Massidda si è avventato contro il senatore Russo, fino ad alzare le mani e a colpirlo. Questo momento di confusione in Aula ha indotto la presidente Mauro a sospendere la seduta per cinque minuti. Dopo la sospensione, la seduta è ripresa come se niente fosse accaduto, semplicemente perché i due senatori in questione si sono dati la mano. Sono ben felice che l'incidente si sia concluso positivamente sul piano personale, ma il problema istituzionale rimane irrisolto. Signora Presidente, colleghe e colleghi, com'è possibile che il Senato della Repubblica italiana possa essere offeso dal sottosegretario Giro senza che ci siano una reazione da parte della Presidenza del Senato e le scuse del Governo? Come è possibile che un senatore possa alzare le mani su un collega senza che ci sia una reazione da parte della Presidenza del Senato? Colleghe e colleghi, dove siamo arrivati? Cosa è diventato il Senato della Repubblica italiana, la Camera alta presieduta dalla seconda carica dello Stato? caso non c'entra un discorso di maggioranza od opposizione: qui è in gioco il rispetto, il prestigio, la dignità dell'istituzione, è in gioco la dignità di ciascun componente di questa Camera. Come possiamo pretendere che le cittadine e i cittadini rispettino le istituzioni, lo Stato, le regole, la semplice educazione, se senatori della Repubblica italiana e membri del Governo si comportano come appena descritto? Presidente, credo che si siano superati tutti i limiti: penso allo spettacolo indecoroso che diamo al pubblico e alle scolaresche che assistono ai lavori di quest'Aula, ad esempio durante le votazioni elettroniche, con i furbi che votano per gli assenti, dimenticando, a mio modo di vedere, che la furbizia è la negazione dell'intelligenza, della buona educazione e della semplice onestà. Signora Presidente, questo mio intervento potrà anche essere deriso e apparire puerile o addirittura patetico. Personalmente, però, mi sono sentito profondamente offeso nella mia funzione di senatore e ritengo che si sentano offese anche le decine di migliaia di cittadini italiani residenti all'estero che con il loro voto mi hanno affidato il compito di rappresentarli con dignità e onore. Presidente, la invito a prendere i giusti provvedimenti affinché siano richiamati i responsabili degli eventi che ho qui ricordato. La prego inoltre di fare in modo che fatti del genere non si ripetano più e che l'Aula del Senato della Repubblica sia veramente, nel comportamento individuale e collettivo, la Camera alta delle istituzioni italiane. Queste considerazioni possono apparire banali; sono invece convinto che siano di fondamentale importanza e che il distacco dei cittadini dalla politica e dalle istituzioni, la maleducazione diffusa in luoghi pubblici, che spesso sfocia nella violenza, siano incoraggiati e quasi legittimati dal comportamento di certi politici e di alcuni parlamentari in particolare. Signora Presidente, non intendo dare lezioni a nessuno; mi creda, non ho questa pretesa. Certi comportamenti, tuttavia, troppo spesso presenti in quest'Aula, sono incompatibili - e per me difficilmente sopportabili - con la semplice ma sana educazione che mi hanno insegnato i miei nonni, contadini abruzzesi, e i miei genitori operai, emigrati in Svizzera.

giustamente, se la prenda solo con un atto che - ripeto - è di reazione. Abbiamo sbagliato a reagire di fronte a certe provocazioni, però non è giusto che la sensibilità

una cronistoria mettendo in chiaro le posizioni di molte persone che abitano nel nostro Paese.

da una parte non tuteliamo la vita nel grembo delle nostre madri, e dall'altra importiamo i giovanotti